avvenuti nella notte tra il 29 e il 31 maggio scorso in quel di Casal Palocco, quartiere periferico di Roma, quando una cinquantina di persone, risultate poi poliziotti in borghese, hanno fatto irruzione in una villetta

La signora, accusata di aver mostrato un passaporto ritenuto falso dai poliziotti presenti, venne trasferita al CIE di Porto Galeria, mentre la figlia venne affidata ai nonni. Nonostante i tentativi, non ci sono state possibilità per gli avvocati di interloquire con la signora. Avendo poi un giudice di pace confermato che il passaporto della signora risultava contraffatto, è scattata una rapidissima procedura che ha portato all'accompagnamento della signora stessa e della figlia all'aeroporto di Ciampino, ove stazionava un aereo privato austriaco, affittato dal Governo kazako, che ha riportato le due donne ad Astana. Nonostante la dimensione dell'operazione e dello sproporzionato numero di agenti intervenuti, pochi sono stati i giornali che hanno dato risalto alla vicenda. Soltanto «La Stampa» di Torino, in data 5 luglio, ha rilanciato il disperato appello del marito della signora. Il signor Mukhtar Ablyazov è uno strenuo oppositore del presidente del Kazakistan Nazarbayev, un vero e proprio dittatore che sembra godere di buone amicizie nel nostro Paese, e forse non soltanto nel nostro Paese. Nello stesso giorno si è avuta notizia del fatto che la sezione speciale del tribunale del riesame di Roma ha riconosciuto che vi sono state gravi violazioni nelle procedure in ordine alle diverse irruzioni della polizia nella casa di Roma in cui, da settembre del 2012, le due donne (una delle quali, lo ripeto, è una ragazzina di sei anni) vivevano. Sappiamo che il presidente Letta ha assicurato - sono parole del Presidente - «una verifica interna agli organi di Governo che ricostruisca i fatti ed evidenzi eventuali profili di criticità». Noi del Movimento 5 Stelle riteniamo si tratti di fatti non gravi, ma gravissimi, e non ci possiamo accontentare di una semplice indagine interna. Qui si parla di una gravissima responsabilità dell'Esecutivo, che ha avallato e appoggiato una vera e propria procedura di sequestro di persona per

e *media* non tenessero sempre in conto il peso dell'ENI o di chissà chi altro, ma cercassero di conoscere e di raccontare verità, anche se scomode per la proprietà, perché per noi del Movimento 5 Stelle i diritti delle persone valgono più delle aziende, pure se italiane.

vorremmo capire bene cosa è successo al volo intercontinentale Mosca-La Paz, all'interno del quale c'era il presidente della Repubblica boliviana Evo Morales. L'aereo è stato bloccato o, meglio, al velivolo non è stato concesso il permesso di sorvolo su alcuni Paesi europei, compresa l'Italia. capisco che stiamo parlando di altro, però chiedo che l'Aula del Senato possa affrontare tale questione che sta provocando le proteste durissime

PSI)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, senatrici e senatori,

ma di una lunga strada che l'Italia ha innanzi a sé. È lecito attendersi che l'inizio della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, previsto per la seconda metà dell'anno 2014, possa vedere l'Italia in una esemplare posizione virtuosa. Purtroppo, per quanto concerne il metodo, troppe volte, in passato, abbiamo preso l'abitudine di recepire le direttive comunitarie solamente all'apertura della procedura di infrazione, per poi essere costretti a legiferare sotto la pressione della necessità e con estrema rapidità,

Appare più che mai necessario imboccare la strada dell'azione e abbandonare quella della pura reazione, provvedendo al puntuale recepimento delle direttive prima dell'apertura

non dover rinunciare ai fondi che ogni infrazione non chiusa ci costa (30-40 milioni di euro, secondo le informazioni da lei rese, signor Ministro); dall'altra parte, corriamo il rischio di dover restituire all'Unione europea 18 miliardi di euro per mancata capacità di spesa sui Fondi strutturali (sul Fondo sociale, sul Fondo per lo sviluppo rurale, e così via).

il successo che ha riportato il Presidente del Consiglio in merito alla chiusura della procedura di infrazione e sui limiti dell'indebitamento, la messa a disposizione di nuovi fondi per l'occupazione e la ricerca e la maggiore flessibilità

del Governo, del Presidente del Consiglio e anche suo, signor Ministro. Siamo sulla strada che ci porta verso gli Stati Uniti d'Europa, e l'Italia è tornata nel girone dei Paesi di serie A. Credo

Cociancich, Giovanni Mauro e Cardinali, e tutti i membri della Commissione per il lavoro svolto e per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra minoranza linguistica

In particolare, vorrei fare riferimento ai risultati positivi che si sono ottenuti su una questione che ci sta particolarmente a cuore e che riguarda tutta la partita dei diritti umani,

europee. Sono stati conseguiti sicuramente risultati importanti per quanto riguarda la questione dei rifugiati, e di questo voglio ringraziare il relatore, il presidente Chiti e il Ministro. modo, la direttiva 2011/36/UE sulla tratta degli esseri umani ci sta particolarmente a cuore perché riguarda in particolare i bambini e le donne.

il nostro Paese, segno anche di modernizzazione e di investimenti futuri, possiamo essere assolutamente ineccepibili.

Signor Presidente, onorevoli senatori, a conclusione dei lavori di Commissione e d'Aula, il giudizio del Gruppo Lega Nord-Autonomie riguardo alla portata politica dei provvedimenti in approvazione non può che essere critico. Signor Ministro, abbiamo certamente apprezzato il suo impegno in Commissione, ma ciò esula dalla valutazione politica complessiva. Cominciamo subito con il chiarire che non siamo per nulla d'accordo con l'affermazione, fatta da alcuni colleghi in discussione generale, secondo cui il nostro Paese prima di chiedere agli altri più Europa dovrebbe chiedere maggiore impegno a se stesso. No, non siamo affatto d'accordo con questa affermazione, anche perché, se è vero, onorevoli senatori, che l'Italia guida da anni la poco invidiabile classifica dei Paesi che applicano di meno o con maggiore ritardo il diritto europeo, è altrettanto vero che è il Paese che si adegua in modo migliore ai doveri, o sarebbe meglio dire ai *diktat*, di Bruxelles. Attenzione però, perché - e lo abbiamo già ribadito eccesso di rigore ed austerità hanno mandato in rosso i conti degli italiani e stanno causando una profonda crisi del *welfare* ed un prossimo annientamento dei servizi pubblici. Agli occhi dell'Europe, dunque, l'Italia appare negligente; al contrario, invece, agli occhi degli italiani, o almeno agli occhi dei più coscienziosi, questo Paese (o quel che ne resta) sembra essere diventato, negli ultimi anni, una serva remissiva e muta di fronte a tutta l'Unione europea: un vero paradosso al quale i cosiddetti europeisti ad oltranza non sanno, o meglio non vogliono, dare risposta Fatto sta che se il rigido rigore che sta contraddistinguendo la politica europea non sarà contrastato con determinazione dal Governo italiano, si avrà come unico e vero risultato quello di allontanare dall'Europa l'Italia reale, quella che lavora e sopporta il peso della burocrazia, scavando un fossato tra l'opinione dei cittadini italiani del Nord in particolare, e le istituzioni politiche europee, come già accaduto in questi ultimi anni. Il sistema Paese non riesce più a reggere il peso della burocrazia ed anche innovazioni regolamentari, potenzialmente positive, rischiano invece di essere percepite, ancorché non lo siano realmente, come dei vincoli insostenibili, illegittimi e addirittura ingiusti. D'altronde, signor Ministro, non possiamo tacere ad esempio come il Trattato di Lisbona, in abbinamento al dannoso sistema Target 2 del 2007, abbiano portato il Paese ad una sudditanza industriale e commerciale in favore della Germania, contribuendo a gonfiare il *deficit* della nostra bilancia commerciale e mettendo in sofferenza, a catena, tutti i settori produttivi e commerciali. Stridono di fronte a questa realtà gli eccessivi atteggiamenti di euroentusiasmo che hanno accompagnato nei giorni scorsi l'ingresso nell'Unione europea della Croazia o, peggio, l'atteggiamento di cieca apertura nei confronti della Turchia. L'applicazione acritica di nuove norme europee rischia di alimentare invece un crescente sentimento antieuropeo. Ultimo esempio è la recente normativa europea che vieta di coltivare, riprodurre e commercializzare semi di ortaggi che non siano stati approvati dalla nascente Agenzia delle varietà vegetali europee; un nuovo divieto che, paradossalmente, mette nell'angolo anche il recente impegno di questo Parlamento per contrastare la diffusione di semi OGM. Si tratta di nuova norma che ingrassa la burocrazia dell'Unione e stacca una nuova cambiale in bianco alle grandi multinazionali, schiacciando gli interessi della nostra gente e perseguendo una inaccettabile e grigia omologazione. dico guai, se l'essenza dell'Unione europea si traduce semplicemente in una normativa che definisce la dimensione del foglio A4. La traduzione grezza dei provvedimenti che quest'Aula si appresta a votare oggi quale sarà? Semplice: nuova burocrazia. Nuovi adempimenti per rendere la vita difficile alla gente, alle imprese, a chi lavora. Oggi l'Europa si è ridotta a un'unione monetaria dominata dalla logica degli Stati e dalla burocrazia; un progetto che sta mostrando di essere fallimentare e che rende ancora più urgente la realizzazione dell'Europa delle Regioni. Sia chiaro, noi non siamo euroscettici, ma è un dato di fatto che questa Europa, così com'è, non risolve i problemi della nostra gente. Sia altrettanto chiaro che la strada per il futuro dell'Europa sarà sempre più in salita se non prevarranno gli interessi dei cittadini su quelli delle *lobby* finanziarie. Signor Ministro, apriamo gli occhi e non lasciamoci imporre dalla burocrazia europea una nefasta omologazione, di fronte alla quale opporsi diventa invece necessario; ne tenga conto il Governo per le azioni future. Ribellarsi di fronte a queste situazioni è un diritto-dovere di un Governo che voglia difendere i propri cittadini. L'impressione, invece, è quella che, ancora una volta, nelle scelte politiche dell'Unione europea, mentre i francesi difendono gli interessi francesi e i tedeschi quelli tedeschi, gli italiani fanno invece gli europei ad oltranza. Al Governo chiediamo quindi un impegno serio e concreto per far valere in Europa le giuste ragioni del Nord produttivo e dell'intero Paese. Tra le questioni sul tavolo a livello europeo spicca certamente quella del contrasto all'immigrazione clandestina e della gestione dei flussi migratori. Su questo fronte chiediamo un impegno forte al Governo nel dare concreto seguito alla risoluzione approvata dal Senato, perché l'Italia non può essere lasciata sola dall'Europa di fronte a questo problema. Anche in questa occasione, lo ribadiamo: attenzione, perché la politica dell'immigrazione incontrollata che viene applicata in Italia finirà per causare problemi al resto dell'Europa, ottenendo come risultato finale un prevedibile isolamento di questo Negli interventi che mi hanno preceduto si è detto che dobbiamo preoccuparci dell'opinione e della credibilità dell'Italia presso gli altri *partner* europei; noi non siamo d'accordo con questa opinione. Noi, signor Ministro, oggi diciamo a lei e al Governo che dovreste invece preoccuparvi di più dell'opinione che i nostri cittadini hanno dell'Europa (*Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, a partire dall'euro, una moneta che doveva fare l'unità politica ed economica europea e che invece sembra sempre più avere fatto gli interessi dei banchieri e la povertà degli italiani. Il sistema economico e finanziario europeo sta di fatto favorendo lo *shopping* a bassi costi da parte di altri Stati a danno delle migliori industrie italiane. Siamo forse ai saldi di fine stagione? Atti di pirateria industriale ne abbiamo poi già denunciati in questa stessa sede. O il Governo si mette seriamente a rinegoziare in Europa vincoli come il Patto di stabilità, oppure questo è un Paese destinato ad essere schiacciato, con un'economia sempre più spiaggiata. Oggi ci troviamo ad approvare quelli che, in grande sintesi, vengono presentati come atti di adeguamento a disposizioni europee, dando per definito che le stesse siano cosa buona e lodevole già solo per il fatto di essere emanazione europea. Ma non è così, onorevoli senatori, non lo è, a partire dal fatto che questi innesti normativi sono invece il frutto di un sistema di potere finanziario e politico lontano dall'Europa dei popoli che invece noi vogliamo. Viviamo in un Paese che resta marginale perfino nelle scelte che decidono il suo futuro. In Italia, oggi, è evanescente il senso dello Stato e delle istituzioni. Non esiste più una lotta visibile per la difesa dello Stato sociale e dei diritti dei lavoratori. *(**Applausi dal azione di giustizia sociale e di rispetto per la dignità della persona. Anche ogni nostro sforzo per rinnovare il Paese in senso federale e per dare risposta alla questione settentrionale, viene addirittura negato in radice, tanto da destra, quanto da sinistra. Onorevoli senatori, questo è lo specchio di un Paese che ha fallito nella propria ragion d'essere, incapace di schierarsi contro lo strapotere delle banche e delle *lobby* di un'Europa che punta ad essere unione bancaria prima che unione di popoli. Come ogni provvedimento, anche quelli che oggi voteremo contengono delle scelte che valgono un voto positivo e delle scelte che valgono un voto negativo. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, signor Ministro, il Gruppo Lega Nord-Autonomie non darà un voto positivo a questi provvedimenti. Intendiamo con questo voto dare invece una reale rappresentanza parlamentare a tutti i nostri concittadini, delusi da un'Europa che ci soffoca con la burocrazia, da un'Europa intenta a perseguire gli interessi della finanza e delle *lobby*, da un'Europa che sta schiacciando l'economia dell'Italia, a partire dalla sua parte più produttiva, il Nord. A questi nostri concittadini, con questo voto, diciamo chiaramente che non tutti i partiti politici sono uguali e non tutti si sono sottomessi all'Europa delle *lobby* e della finanza. La Lega Nord, che fonda la propria storia nella difesa delle autonomie e delle identità locali, farà una dura opposizione all'Europa della finanza e delle banche. Cosa va fatto lo abbiamo detto; cosa non va più fatto lo abbiamo chiarito. Ora sta a voi, Governo, dimostrare in tema di politica europea di essere all'altezza con le responsabilità che vi siete presi. Chiudendo, al Governo diciamo in maniera chiara:

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto desidero ringraziare il presidente Chiti, i relatori ed il Governo per il lavoro fatto e che avrà il nostro voto favorevole. con la legge n. 234 del 2012 si apre una stagione nuova nelle procedure legislative della legislazione europea, che è riconnessa all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in particolare, ai nuovi poteri di intervento del Parlamento nel processo decisionale europeo, nonché all'esigenza di una più tempestiva attuazione degli obblighi europei. In realtà, il provvedimento appare volto primariamente a porre rimedio a lacune e carenze strutturali della partecipazione del sistema Paese al processo di formazione e di attuazione delle politiche europee che si erano già manifestate ben prima dell'adozione del nuovo Trattato e si erano acuite con la progressiva evoluzione costituzionale europea. Innestandosi su questi processi già avviati, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha contribuito ad accrescere la consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza di un adeguamento delle procedure nazionali, sia in relazione alle nuove prerogative espressamente conferite ai Parlamenti nazionali, sia indirettamente in funzione del nuovo assetto costituzionale dell'Unione europea da esso determinato e delle stesse innovazioni introdotte in altri ordinamenti in relazione all'attuazione del Trattato stesso. Un ruolo non secondario nella predisposizione della legge è stato esercitato, poi, dalle dinamiche istituzionali e politiche sviluppatesi a livello europeo a seguito dell'acuirsi della crisi economica e finanziaria. La costruzione - tuttora in corso - di un nuovo sistema di *governance* economica, elaborato ed attuato mediante strumenti e procedure prettamente intergovernativi, ha reso infatti urgente, in Italia come in altri Stati membri, la definizione di appositi strumenti di controllo parlamentare. In coerenza con questa lettura, si è proceduto all'adozione di disposizioni costituzionali, legislative e regolamentari atte ad un più generale consolidamento del raccordo tra Parlamento e Governo. Questa è quindi l'occasione per riflettere sui nuovi strumenti offerti dalla legge n. 234, che è una delle vere grandi leggi di riforma della scorsa legislatura nel nostro Paese. Infatti, se da un lato si celebra con enfasi l'approvazione del Trattato di Lisbona, dall'altro matura sempre più la consapevolezza che la vera sfida stia nel verificare che nella pratica i singoli Stati accettino pienamente la parziale cessione di sovranità a favore dell'autonomia europea che lo stesso Trattato prevede, nel rispetto del principio di sussidiarietà. L'obiettivo politico principale che ci si era posti con il Trattato era proprio quello di colmare un *deficit* di rappresentanza che aveva reso la burocrazia dell'Unione europea sempre più distante e percepita addirittura come ostile dai cittadini. Il pericolo maggiore per il processo d'integrazione europea era ed è individuabile proprio nella diffidenza verso le istituzioni di Bruxelles, alimentata in questi anni da schieramenti populisti e xenofobi, fautori della supremazia delle Nazioni su ogni organismo sovranazionale e addirittura nella reclusione rassicurante delle aspirazioni delle comunità locali nelle cosiddette piccole patrie. Non ha proprio senso una contrapposizione tra l'Europa Oggi questo pericoloso processo di disgregazione rischia di essere alimentato dall'onda dello *tsunami* che ha investito l'economia e i mercati finanziari. Il ripiegamento su logiche strettamente nazionali, che hanno pesato quando bisognava prendere decisioni importanti e rapide in favore di Paesi in difficoltà (vedi la Grecia), è un comportamento che spesso non ha pagato. È illusorio infatti pensare che qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, a partire dai più grandi, possa far valere i propri interessi nazionali al di fuori di uno sforzo congiunto europeo. La realtà internazionale è talmente cambiata che non si vede come alcuno dei singoli Paesi possa recuperare un suo ruolo autonomo e distinto per reagire con le sue forze alle sfide della globalizzazione; ciò vale per la lotta all'inquinamento, la criminalità organizzata, il terrorismo, una nuova *governance* mondiale monetaria anche relativa all'apertura dei nuovi mercati, a cooperazione internazionale allo sviluppo. È in questo quadro che occorre inserire un nuovo protagonismo italiano in Europa, che richiede innanzitutto fiducia in se stessi, evitando le solite litanie piagnone che riscontriamo in chi preferisce continuare a vedere le pagliuzze negli occhi altrui ma non le travi nei Per troppo a molti è apparsa una perdita di tempo dibattere sulle questioni degli assetti istituzionali piuttosto che concentrarsi sulle decisioni da prendere per affrontare la crisi economica; questo perché ai più sfuggiva che proprio le insufficienze delle istituzioni europee hanno da sempre limitato gravemente la capacità dell'Europa di agire unitariamente e di far sentire il suo peso sullo scenario mondiale. La crisi economica ci ha aiutato in questa direzione. Oggi è maturata in Europa la consapevolezza, grazie anche all'azione del Governo Monti prima e dell'Esecutivo Letta poi, che una politica incentrata esclusivamente sull'autorità e sull'austerità di bilancio è insufficiente ma necessaria e va accompagnata con le pratiche per la crescita che richiedono la capacità di cogliere le opportunità che la globalizzazione ci offre. Il Governo italiano oggi ha l'importante compito di proseguire un cambiamento di rotta, avviato dal Governo Monti in queste scelte, e di indicare un percorso di ripresa che sia condiviso e compreso dai cittadini. Bisogna avere l'ambizione di guardare alla ripresa, puntando su strumenti in grado di garantire la crescita senza dilatare il debito.

di un più grande potere legislativo europeo, dobbiamo sentirci legislatori nazionali all'interno di questo processo. La legge n. 234 ci ha spinto in questa direzione e noi vogliamo essere coerenti rispetto a questo grande risultato che oggi otteniamo

che ha determinato l'adozione dei principali atti relativi alla partecipazione del nostro Paese alla formazione e all'attuazione della normativa europea, secondo quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. In particolare, mi sia consentita una breve digressione sulla legge stessa. Come è noto questa è la novità che abbiamo dovuto tutti tutti affrontare in questa legislatura. All'articolo 30 di questa legge si definiscono sia la legge di delegazione europea, nella fattispecie il disegno di legge n. 587,

dei decreti legislativi di recepimento di direttive europee. In sostanza, con questa legge il Governo chiede al Parlamento la delega a legiferare al suo posto, seppure per il nobile e necessario scopo di recepire le direttive europee. Ripeto: il Governo chiede al Parlamento la delega a legiferare al suo posto. Questa modalità, però, stride fortemente con la troppo spesso celebrata centralità del Parlamento. È quindi un altro esempio dello svuotamento del ruolo del Parlamento, sempre sempre più semplice ratificatore di decisioni prese dal Governo. Ciò dimostra, inoltre, che i vertici che comandano il modello unico non si fidano neanche dei loro stessi parlamentari, ai quali si chiede solo di confermare, ratificare e convalidare decisioni prese dall'Esecutivo, o forse solo dai vertici dei partiti del modello unico. Tutto questo a noi del Movimento 5 Stelle Preferiremmo un ruolo più attivo del Parlamento anche in queste occasioni, che sembrano di mero, passivo recepimento di direttive dell'Unione europea per le quali invece il Parlamento può e deve dire la sua imponendo, secondo i limiti previsti dalla legge n. criteri e vincoli corrispondenti ai veri *desiderata* dei cittadini italiani. Alternativamente, il Parlamento si dovrebbe attivare in autonomia per recepire le opportune direttive dell'Unione europea, ma soprattutto dovrebbe forse influenzare di più, insieme agli altri Parlamenti nazionali, l'attività legislativa dell'Unione europea, alzando così il livello di democraticità delle istituzioni europee. Ma forse questo poco interessa. In quest'ottica, non vogliamo essere come le altre forze politiche, che riteniamo troppo spesso supinamente euro-acritiche, si adagiano, si crogiolano e si compiacciono in un ripetuto e quasi quasi agiografico riferimento all'Europa e ai futuribili, non si sa quando, Stati Uniti d'Europa.

al condizionale - sarebbe sicuramente favorevole, essendo questo l'atto contenente tutte quelle norme diverse dalle deleghe necessarie ai fini dell'adempimento di obblighi europei e finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea stessa. Come illustrato dal relatore, si tratta di direttive importanti, utili, ad esempio, a garantire la libera circolazione dei cittadini all'interno dell'Unione, oppure il libero accesso alla professione in qualsiasi suo Stato. Questo nel Questo nel Capo I della legge europea, che prosegue con gli articoli del Capo II, riguardanti la fiscalità, del Capo III, riguardanti il lavoro, del Capo IV, riguardanti la sanità pubblica, del Capo V, riguardanti l'ambiente, del Capo VI,

alcuni dei criteri presenti in questo articolo, noi del Movimento lo riteniamo insufficiente, in quanto impone criteri di recepimento che a molti di noi paiono non idonei a limitare le sofferenze degli animali oggetto di sperimentazione e e sicuramente non in grado di garantire i necessari controlli e le doverose ispezioni nelle strutture ove questa pratica, purtroppo, avrà comunque luogo; non rappresentano inoltre un reale impulso alla ricerca e all'applicazione di metodi alternativi all'utilizzo di animali nelle fasi di studio e di analisi di un nuovo farmaco. Ci rammarichiamo perciò dell'assoluta insensibilità e indisponibilità da parte delle altre forze politiche e soprattutto del Ministero della salute evidenziata dal non aver voluto recepire positivamente i nostri emendamenti all'articolo 12 (inizialmente articolo 9), volti a migliorare in fase ascendente nella Commissione preposta (la 14ª), questa norma. Pertanto, questi emendamenti, in combinato disposto con l'articolo 12, avrebbero completato un quadro legislativo che avremmo considerato di reale, concreta ed effettiva tutela per le specie animali.

scientifica alle missioni internazionali, dai bilanci degli Stati al commercio di prodotti tecnologici, per passare a norme finanziarie. Evidentemente, tutta materia che può rientrare, per omogeneità, nello stesso provvedimento. Benissimo, tutto questo questo permette al Movimento, in maniera assolutamente chiara e politicamente forte, di lasciare a tutti i senatori del Gruppo libertà di voto; non perché non ci vogliamo prendere le nostre responsabilità, perché noi le responsabilità ce le prendiamo, ma perché voi, signori del Governo, e comunque signori del modello unico, avete il coraggio di imporre una logica per cui o si prende tutto oppure non si deve prendere niente. Vorremmo che vi fosse - e questa ci sembra democrazia - la possibilità di ragionare pacatamente su singoli temi, su singoli provvedimenti, su cui il Movimento 5 Stelle darà certamente il suo contributo. Non è affatto vero, infatti, che noi siamo soltanto quelli della protesta; noi siamo anche quelli della proposta e in Commissione abbiamo cercato di farvelo capire in tanti modi. Ma evidentemente i tempi che imperiosamente voi dettate al dibattito parlamentare (altrimenti non si fa in tempo ad approvare) sono quelli che vogliono far passare insieme al provvedimento intelligente anche quello su cui si potrebbe intervenire per rettificare. Il Movimento 5 Stelle su questo non ci sta. Per questo tutti quanti noi, con senso di responsabilità, accettiamo la logica della libertà di voto e richiamiamo per l'ennesima volta per mezzo di un Ministro - che è qui presente - l'impegno che aveva assunto lo stesso presidente del Consiglio Letta: cerchiamo di farla finita con i provvedimenti *omnibus*. Permettiamo a tutti i senatori, a tutti i parlamentari - perché anche in altri Gruppi ci sono singoli parlamentari che hanno le nostre stesse difficoltà

il Presidente, tutti i componenti della 14a Commissione del Senato e, in particolare, i relatori che, con un lavoro alacre e diuturno, hanno dovuto elaborare e codificare gli emendamenti alle due leggi, che si parano questa sera innanzi a noi per l'approvazione a causa dell'interruzione anticipata della XVI legislatura che vengono, quindi, a riempire il vuoto determinato dalla mancata approvazione delle leggi comunitarie 2011 e 2012. Questi provvedimenti del Governo credo vadano nella direzione di recepire le direttive comunitarie attraverso la delega legislativa; non potrebbe che essere così, atteso che si tratta di adeguare, correggere e integrare la legislazione nazionale di sopperire ad eventuali inadempienze da parte dell'Italia nel far proprie le disposizioni europee, soprattutto nell'intento di evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione ai danni della nostra Nazione. È appena il caso di ricordare che ogni ulteriore indugio nell'approfondimento dei temi legati a questi disegni di legge esporrebbe il Governo a gravi difficoltà circa l'emanazione e l'adozione di decreti delegati in materia di particolare rilevanza. La legge di delegazione europea attiene *in primis* al recepimento di specifiche direttive in tema di inquinamento ambientale. Altri aspetti significativi, a mio parere, riguardano la contabilità e la finanza pubblica e sono oggetto di interventi migliorativi dell'impalco legislativo, con particolare riferimento ad una nuova disciplina dell'IVA, nonché alla riaffermazione - ahinoi - del principio di pareggio di bilancio. senza sottacere le profonde modifiche proposte per la gestione dei fondi alternativi, al fine di evitare i rischi che hanno accompagnato le fasi più acute della crisi finanziaria

è opportuno ricordare altre importanti innovazioni presenti in questo disegno di legge, nel campo del commercio, della sanità, dei diritti civili per gli stranieri. Un ulteriore passo avanti è costituito dal recepimento, nella legge europea, delle normative che pongono riparo alla disattesa applicazione del diritto comunitario, lamentata da cittadini ed imprese, molte volte costretti a ricorrere contro il mancato rispetto del loro buon diritto. Per motivi di tempo occorre limitarsi a riaffermare l'incisività delle iniziative da assumere in materia di politica ambientale, così come scaturiscono dall'attuazione della direttiva n. 75 del 2010 dell'Unione e per quanto riferibile alla gestione dei rifiuti industriali, ma anche delle autorizzazioni, dei controlli e delle sanzioni nel campo dei rifiuti in genere. Questo al fine di evitare, attraverso un efficace controllo delle autorizzazioni, il riproporsi di situazioni di devastanti danni ambientali, che assumono connotazioni di particolare gravità nel Mezzogiorno; e sono ancora recenti le immagini di Napoli invasa dai rifiuti e di una Campania e di una Sicilia spesso collassata per fenomeni che sono certo a monte e per la mancata attuazione di un'avanzata politica di trattamento di rifiuti stessi, ma anche perché spesso la nostra legislazione è stata lacunosa sotto il profilo dell'incisività e della forza coercitiva nei confronti dei dei demagoghi che, a vario livello, abbiamo trovato sia nelle amministrazioni provinciali, che nelle stesse amministrazioni regionali. In questo disegno di legge, in campo finanziario assume risalto l'urgente implementazione dei vigenti dispositivi di legge, collegandoli ad un inevitabile adeguamento dell'IVA alla legislazione europea.

inoltre l'adozione delle direttive europee in campo sanitario; vi è infatti la necessità di indirizzare la riforma delle regole sulla farmacovigilanza sancite dalla direttiva n. 26 del 2012. In tema di salute pubblica vanno anche posti nel dovuto risalto i diritti sanciti per i pazienti frontalieri negli Stati aderenti all'Unione europea, tenuto conto dell'imminente adozione della direttiva n. 24 del 9 marzo 2011, cosi come assume rilievo l'intensificazione del controllo delle pratiche di sperimentazione in campo animale.

nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti sia dai trattati Maastricht che da quelli di Lisbona. quindi il nostro voto favorevole, constatata l'osservanza della regolarità tecnica in ordine agli oneri finanziari derivanti dall'adozione dei provvedimenti in oggetto e preso atto del rispetto del principio di sussidiarietà. La puntuale affermazione di questo principio nella legge europea si rileva essenziale ai fini di un corretto rapporto tra Stato e società, che - mi consentirete di ricordarlo - deve essere sempre più ampliato in quelle società aperte ed evolute, ove il diritto e il dovere di organizzare le forme di convivenza sul piano sociale e civile spetta ad associazioni, sindacati, a privati cittadini, affinché siano garantite ed ampliate, in buona sostanza, attraverso l'applicazione di tale principio, le libertà le libertà negative, come le chiamava *Isaiah Berlin*. Queste libertà sono l'aspetto saliente della libertà del cittadino stesso in quanto appartengono alla sfera dei diritti che non sono nella disponibilità di alcun potere politico, giudiziario o istituzionale. Per quanto concerne, quindi, il Popolo della Libertà siamo convinti di dover dare il nostro assenso e il nostro voto favorevole a questa legge.

del Ppartito Democratico voterà a favore di questo pacchetto di norme e documenti di armonizzazione della legislazione nazionale con quella europea, nonché di valutazione e di indirizzo alle politiche dell'Unione europea, con la consapevolezza che in questo momento i temi che ci legano all'Europa, come è stato ricordato recentemente anche dal Presidente della Repubblica e dal nostro Presidente del Consiglio, devono rappresentare per l'Italia la priorità e l'orizzonte di azione sia del Governo che del Parlamento. Il lavoro, proficuo, compiuto dalla Commissione e dall'Aula va appunto nella direzione di superare la logica dei temi europei intesi come separati e estranei al nostro ordinamento, puntando, invece, ad inserire appieno nella politica nazionale e nel processo legislativo che la informa il rapporto tra Stato ed Unione europea come costitutivo. L'Unione europea costituisce a tutti gli effetti un'ulteriore sede legislativa, intimamente legata all'ordinamento interno italiano, cui copartecipiamo come soggetti consenzienti nell'elaborazione delle norme. Il tema è, appunto, quello della consapevolezza e della partecipazione attiva: lo è per il Parlamento quanto per i cittadini italiani. In una fase politica ed economica di grande difficoltà, il sentimento nazionale ed il discorso politico rischiano di sclerotizzarsi in una falsa dialettica tra pro e Siamo oltre: non dobbiamo più scegliere l'Europa, l'abbiamo fatto molti decenni fa; è una scelta costitutiva, irrinunciabile politicamente ed economicamente, soprattutto nella crisi. Dipende solo da noi uscire dalla logica della resistenza, dell'adeguamento passivo e burocratico alla legislazione europea e passare alla partecipazione attiva politica alla costruzione normativa. Dobbiamo passare dalla logica del negoziato, tipicamente intergovernativa, a quella della costruzione del processo democratico europeo. Il Parlamento può e deve fornire - lo dico al senatore Morra - il proprio contributo in maniera determinante, avvalendosi dei mezzi che sono, da ultimo, messi a disposizione dall'innovazione normativa contenuta nella legge n. 234 del 2012. n. 234 del 2012. Anche grazie a questa legge e al lavoro del Parlamento, dopo due anni di blocco legislativo, l'obiettivo prioritario del nostro lavoro in Commissione e in Aula è stato, infatti, quello di procedere il più speditamente possibile all'esame dei provvedimenti per contribuire sensibilmente a ridurre il numero delle infrazioni, che costituiscono un peso economico non sopportabile nella fase attuale e un peso politico perché pregiudicano la stessa credibilità dell'Italia nelle sedi europee. Abbiamo cercato di farlo, appunto, in modo non burocratico, ma considerando e contemperando l'istanza comunitaria insieme alle istanze nazionali che sono state presentate alla nostra attenzione. Mi riferisco sia a quelle più datate trascinate dalla mancata approvazione per per un biennio delle leggi comunitarie, sia a quelle emerse recentemente su temi estremamente rilevanti, quali, ad esempio, il regolamento europeo in materia di IVA, le questioni connesse alla tutela ambientale, la spinosa questione del recupero degli aiuti dati dal nostro Paese alle imprese e ai cittadini colpiti da calamità naturali; a tutte queste, con il nostro lavoro in Commissione, abbiamo tentato di dare risposte adeguate e in tempi brevi. la legge europea risente maggiormente del ritardo ed è, conseguentemente, più ricca di norme. Nell'azione di contenimento e prevenzione delle infrazioni abbiamo cercato di tenere l'orizzonte dei diritti, ragione della Costituzione europea, e di tenere in primo piano l'interesse generale dei cittadini anche nell'accettazione dei divieti. In questo senso vanno le disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone, nonché quelle riguardanti l'ambiente, con puntuali modifiche alla legislazione italiana in materia di tutela delle acque, di valutazione integrata ambientale, di gestione dei rifiuti e di tutela risarcitoria contro i danni ambientali. Laddove sono in gioco interessi contrapposti, abbiamo cercato mediazioni ragionevoli e - dove possibili - al rialzo. È il caso, ad esempio, delle guide turistiche, dove il giusto principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati dell'Unione è stato temperato dalla previsione, per il nostro Paese, di richiedere una speciale autorizzazione per i siti di particolare interesse storico ed artistico, che sono uno degli elementi costitutivi per il rilancio economico del nostro Paese. L'abrogazione dell'articolo 34, in materia di utilizzo dei brevetti di *design* industriale non protetti, e lo stralcio dell'*ex* articolo 33, in materia di agevolazioni fiscali e contributive riconosciute per i terremoti che hanno colpito il nostro Paese dal 1997 al 2009, danno conto della necessità di non riversare sui cittadini e le imprese le contraddizioni di decisioni prese in fasi politiche ed economiche anche molto lontane nel tempo e di trovare, con l'approfondimento e il tempo necessari, soluzioni in grado di garantire equità e sostenibilità. Anche nel disegno di legge di delegazione europea 2013 ci sono buone novità. Tra queste, vorrei ricordare nella complessa vicenda che riguarda i regolamenti in materia di IVA, abbiamo previsto, con l'approvazione di un emendamento, che sia tenuta in considerazione la peculiarità, tutta italiana, dello svolgimento in sussidiarietà di prestazioni sociosanitarie da parte di soggetti della cooperazione sociale, in grado di sostenere un *welfare*, diversamente già fortemente ridotto e penalizzato dalle necessità di contenimento della spesa pubblica. Un buon lavoro è stato svolto anche nella definizione di adeguati criteri di delega per l'attuazione della direttiva europea in materia di riconoscimento dei diritti dei beneficiari di protezione internazionale. così testimoniata la volontà del Paese di dotarsi di una legislazione che, secondo lo spirito della Convenzione di Ginevra, possa assistere e proteggere i rifugiati presenti sul nostro territorio, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati e alle vittime di tratta. Infine, mi sembra importante rilevare il buon compromesso al rialzo ottenuto in Commissione per quanto concerne la delicatissima questione della sperimentazione animale, che, nel garantire quanto disposto in sede europea (quindi nel pieno rispetto della direttiva europea), fa salve le istanze radicate nel Paese che mirano ad una maggiore tutela e protezione degli animali utilizzati a fini di ricerca. Abbiamo svolto questo lavoro mentre il nostro Governo sedeva al tavolo del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno: i risultati ottenuti ci danno speranza che, nel prossimo Quadro finanziario 2014-2020, le politiche relative alla crescita e all'occupazione, gli aspetti di politica estera e di vicinato e gli orientamenti espressi nelle risoluzioni che proponiamo oggi al voto dell'Aula siano pienamente assunti come prospettiva di sviluppo. È fondamentale, infatti, che continui l'impegno del Governo, pienamente sostenuto dal Parlamento, nella promozione di politiche dirette ad affiancare, al rigore fiscale, misure in grado di stimolare la crescita e l'occupazione. Tra queste, l'emissione di titoli obbligazionari europei da destinare al finanziamento di investimenti di interesse europeo. In questo senso, accogliamo con soddisfazione l'apertura del presidente Barroso, a «deviazioni temporanee» dagli obiettivi di bilancio previsti dal Patto di stabilità in caso di investimenti pubblici legati a misure per favorire la crescita, per Paesi, come l'Italia, che hanno i conti in ordine perché hanno fatto i compiti. Il cambiamento di prospettiva che abbiamo auspicato e per cui ci siamo battuti sembra finalmente affacciarsi: consentire investimenti pubblici produttivi, cofinanziati dall'Unione europea, capaci di far ripartire il sistema Paese, uscendo dalla fase più dura della crisi economica di questi anni è fondamentale per raggiungere l'obiettivo di rilanciare il Paese e anche di conseguire il pareggio di bilancio di medio termine. Gli italiani, che hanno fatto i conti con il rigore del bilancio, possono pretendere che si investa sulla loro serietà e sulla capacità del sistema Paese di rimettersi rimettersi in moto. Possono pretendere che diventino concrete le ragioni per le quali stare in Europa è ancora una volta un'opportunità e, prima di tutto, un'opportunità che occorre saper sfruttare.

apre una nuova finestra"). Prima di passare alle votazioni finali, avverto che, con riguardo ai disegni di legge al nostro esame, sono state presentate due distinte proposte di coordinamento

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012*** Il relatore, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

Finalmente essi sono superati, e con il provvedimento oggi al nostro esame ratifichiamo una Convenzione tra la nostra Repubblica e quella di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. Dicevo che si tratta di normalizzare i rapporti tra i nostri Paesi dopo tante battute d'arresto e tanti ostacoli che ci sono stati in questi anni. La Camera ha approvato recentemente il disegno

La nuova formulazione del testo mira a rendere più penetrante la collaborazione in campo fiscale, prevedendo che lo Stato oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Lo Stato richiesto non potrà dunque rifiutare di fornire informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da soggetti similari. Dunque, onorevoli colleghi, questo comporta, come è a tutti chiaro, una forte riduzione della portata del segreto bancario. Una clausola esclude, peraltro, alcuni benefici reciproci qualora lo scambio di informazioni non sia adeguatamente applicato. Capite che per San Marino questo significa il rientro a pieno titolo nella *white list* delle organizzazioni internazionali; questa nuova legittimazione produrrà benefici a San Marino, ma anche al tessuto produttivo in particolare delle Marche e dell'Emilia-Romagna, facilitando gli investimenti per infrastrutture e imprese che operano in quel territorio. Sul tema della collaborazione e della trasparenza ci sono i benefici maggiori per l'Italia nel suo complesso; per dirla con una battuta: quello che discutiamo oggi è un accordo per evitare le doppie imposizioni fiscali, ma contiene anche strumenti essenziali per evitare che di imposizioni fiscali invece di due non ce ne sia nemmeno una. La questione è dunque di giustizia sociale, tema fondamentale nel rapporto tra Stato e cittadini. L'evasione fiscale è un fenomeno intollerabile che va colpito con accordi come questo, soprattutto in periodo di crisi economica e di tanti sacrifici per le famiglie. Se n'è accorta anche l'Europa; infatti, al Vertice europeo di fine maggio si è parlato di questi temi e l'Unione si è impegnata a modificare la direttiva sulla cooperazione amministrativa tra diversi Stati per ricomprendere nello scambio automatico di informazioni tutte le forme di reddito, e si è anche impegnata a sostenere questo principio in tutte le sedi internazionali, oltre che bilaterali. Sottolineo, per concludere, che la Convenzione permette anche di avviare a soluzione l'annosa questione dei lavoratori transfrontalieri. A San Marino lavorano più di 6.000 italiani, che rappresentano il 30 per cento della forza complessiva; questi lavoratori sono sottoposti a una situazione fiscale intollerabile, anche per l'imposta introdotta nel 2011 dalla Repubblica del Titano. La Convenzione precisa che i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza. L'Unione dovrà definire le modalità di tassazione di questi redditi. Mi auguro che questa legge venga approvata rapidamente, anche perché il Governo ha già assunto un impegno formale in tal senso.

la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali e il relativo Protocollo di modifica sono

La ratifica del Protocollo comporta l'automatica operatività anche degli accordi siglati nel 2002, sulla cooperazione economica, e nel 2009, sulla cooperazione in materia finanziaria, che non sono mai entrati in vigore essendo vincolati all'ultimo tassello riguardante le doppie imposizioni. i temi di maggiore rilevanza politica definiti mediante l'accordo sono lo scambio di informazioni e l'introduzione del reato di evasione fiscale da parte di San Marino. In particolare, i reati di dichiarazione fraudolenta e di omessa dichiarazione saranno introdotti con la riforma fiscale in discussione

Il cardine del nuovo impianto normativo è l'impossibilità di apporre il segreto bancario alla richiesta di scambio di informazioni. questo trattato, che all'Italia costa più di 3 milioni di euro all'anno, viene siglato a vantaggio di San Marino. All'Italia viene garantito uno scambio di informazioni utili per cercare di evitare e reprimere l'elusione e l'evasione fiscale, da sempre una piaga nei rapporti tra i due Stati.

ad adottare le opportune iniziative volte a monitorare: il traffico di capitali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino; quali e quante sono le società costituite nella Repubblica di San Marino che percepiscono utili o dividendi o canoni o interessi di origine italiana; quali e quante saranno le nuove società che si costituiranno nella Repubblica di San Marino nell'arco di 36 mesi e che percepiranno utili o dividendi o canoni o interessi di origine italiana; quali e quante saranno le società costituite nella Repubblica di San Marino che percepiranno utili o dividendi o canoni o interessi di origine italiana, che a loro volta siano partecipate o

è stato appena illustrato il disegno di legge all'esame dell'Aula concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. Poiché si parla tanto di imposizioni in materia di imposte sul reddito tra l'Italia e uno Stato estero a noi confinante, vorrei mettere in evidenza una criticità che riguarda una specifica categoria di lavoratori e lavoratrici che varcano tutti i giorni i confini italiani per andare a lavorare all'estero. Sono i lavoratori frontalieri, e forse non tutti sanno che oggi è l'ultimo giorno che hanno a disposizione per pagare l'imponibile IRPEF. Signori colleghi, intendiamoci, loro sono i primi che vogliono pagare le tasse, ma in sostanza l'inasprimento fiscale prodotto dalla nuova disposizione introdotta con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012),

sia per l'anno in corso, quindi per il 2013, che per il 2014, senza tener conto della franchigia fiscale di 6.700 euro, prorogata con la stessa legge di stabilità 2013. Signor rappresentante del Governo, è evidente che tale tipo di imposizione fiscale è iniqua, discriminatoria e fortemente penalizzante per una categoria di lavoratori e lavoratrici che da sempre è considerata una risorsa per il nostro Paese, in quanto "importatori" di conoscenze in grado di produrre redditi assoggettabili a tassazione in Italia, anche in considerazione del difficile periodo di crisi economica che il nostro Paese sta attraversando. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, stiamo parlando di oltre 60.000 lavoratori che varcano i confini con la Svizzera, di 1.500 con la Francia, di 3.700 con il Principato di Monaco, di 5.400 con San Marino, 1.894 con la Città del Vaticano, di 1.000 con l'Austria e infine di 1.500 con la Slovenia. Come si può capire, sono molte le famiglie coinvolte. Signor Presidente, questo è un problema che si presenta ad ogni scadenza di pagamento dell'IRPEF, e ogni anno viene rimandata una possibile soluzione all'anno successivo, mantenendo così in ansia decine di famiglie italiane. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, poiché mi è stato detto che non ci sono stati i cosiddetti tempi tecnici per rispondere ad una specifica interrogazione da me presentata, e cofirmata dal senatore Micheloni, su tale argomento, mi sembra d'obbligo riparare a questa confusione fiscale, e mi auguro che per il mese di novembre, al momento del saldo, questa categoria di lavoratori risulti a credito e non debba pagare più nulla per quanto riguarda la seconda rata di acconto. Confidando nel buon lavoro di questo Governo e di questo Parlamento, questo sarebbe il momento per definire uno statuto per risolvere una volta per tutte tale contenzioso con i lavoratori frontalieri. Vi ringrazio per avermi ascoltato.

Signor Presidente, svolgo un breve intervento perché nella prima votazione il senatore De Siano ha votato per la senatrice Longo, che non è presente. Prego cortesemente i colleghi di votare regolarmente.

Signor Presidente, i contenuti di questo provvedimento sono stati bene illustrati dal collega relatore, presidente Casini, e negli interventi dei colleghi, in particolare della Commissione esteri. Credo che non sfugga a nessuno la necessità di approvare approvare questo provvedimento in tempi celeri e capisco anche che lo stesso debba fare io: quindi, mi limito esclusivamente a confermare quanto detto in Commissione circa la bontà del contenuto di questo provvedimento e a dichiarare il voto favorevole della Lega Nord.

Signor Presidente, il Gruppo di Scelta Civica per l'Italia esprime voto favorevole a questa ratifica, esame dopo un confronto duro, aspro, ma costruttivo con la Repubblica di San Marino. In questo confronto sono stati superati parecchi ostacoli, ma si è operato all'interno di una cornice che, come è stato detto, è quella che è stata individuata nell'ambito OCSE. Diamo così un apporto concreto all'applicazione delle migliori pratiche e soprattutto di una più forte trasparenza in campo fiscale. Viene ridotta la portata del segreto bancario e San Marino può - come ci veniva qui ricordato dal relatore - rientrare a pieno titolo nella *white list* internazionale. Ma anche l'Italia riceve un vantaggio: questo vantaggio è evitare le doppie imposizioni fiscali, con conseguente beneficio delle imprese delle Marche e dell'Emilia-Romagna.

Signor Presidente, la Convenzione sulle doppie imposizioni fiscali con la Repubblica di San Marino affronta anche la questione della doppia tassazione. Pagare le tasse, noi lo sappiamo ormai bene, è giusto e necessario, anche se spesso è doloroso; pagarle due volte ed ingiustificatamente diventa insopportabile. Questo tipo di accordi bilaterali predispongono argini e vigilanza soprattutto alle frodi; con riguardo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, di cui il

la collaborazione fattiva tra i due Paesi. Infatti, disciplina, tra l'altro, l'importante trattamento fiscale dei redditi da lavoro di circa 6.000 lavoratori frontalieri italiani a San Marino

Le questioni che hanno riguardato i contenuti, oggi risolti all'interno della Convenzione, sono state le cause principali che hanno reso complicati, a volte nascosti e quanto meno difficoltosi, gli scambi finanziari, di merci e di prestazioni tra i due Paesi, Paesi, a dispetto delle profonde affinità culturali, storiche, ma anche economiche e sociali, tra i cittadini in questi residenti. Le questioni che riguardano, da un lato, il rischio di duplicazione della tassazione sui redditi prodotti e percepiti dai non residenti e, dall'altro, il pericolo di frodi fiscali trovano nel testo oggi in discussione soluzioni forti, che penetrano in modo profondo negli ordinamenti dei due Paesi e che hanno tenuto conto della dimensione qualitativa e quantitativa delle relazioni tra gli stessi. Gli scambi commerciali tra Italia e San Marino ammontano oggi a 4,5 miliardi di euro ogni giorno - come avete sentito - più di 5.000 lavoratori, residenti in Italia, prestano la propria opera all'interno dei confini di San Marino, rappresentando il 40 per cento della forza lavoro del settore privato. Gli scambi sicuramente si sono intensificati anche come risultato della scelta molto netta da parte della Repubblica di San Marino di puntare sullo sviluppo dell'economia reale, che ha richiamato dall'Italia forza lavoro, con una progressiva contrazione dell'attività del settore creditizio. Di qui l'avvio di una serie di riforme volte a far uscire il Paese dalla *black list* delle organizzazioni internazionali. Nel corso degli ultimi anni la Repubblica di San Marino ha infatti assunto, anche in modo formale, l'impegno di adeguarsi ai princìpi OCSE in materia di concorrenza e trasparenza bancaria, eliminando gli spazi giuridici e le forme societarie che sono state la causa di effetti distorsivi dei rapporti e che rappresentavano di fatto la barriera più rilevante allo sviluppo delle imprese. A tal fine, l'accordo, che prevede l'eliminazione delle società anonime, il contrasto agli illeciti tributari e una notevole apertura in materia di rogatoria, amplia di fatto la collaborazione in campo fiscale, riducendo notevolmente gli spazi del segreto bancario. Stabilisce infatti lo scambio automatico delle informazioni relative a tutte le forme di reddito e diventa quell'efficace strumento contro l'elusione e l'evasione fiscale che il nostro Paese sta cercando di costruire e su cui anche l'Unione europea sta lavorando per estenderlo alle sedi internazionali e ai rapporti bilaterali. Pone inoltre a soluzione il rischio pieno di potenziale iniquità della doppia tassazione dei redditi e, in particolare, di quelli percepiti dai tanti lavoratori transfrontalieri. Si stabilisce infatti che i redditi saranno definitivamente tassati nel Paese di residenza del percepiente. Le nuove regole bilaterali tra Italia e San Marino in campo fiscale aprono quindi una nuova strada per la collaborazione e la cooperazione dei due Paesi, Paesi, fondata di fatto su una integrazione più spinta tra i cittadini e su un netto rafforzamento delle dinamiche economiche, che assegnano all'Italia un ruolo estremamente rilevante, visto che è l'unico Paese confinante e il *partner* economico più rilevante. Il voto di oggi, dopo quello favorevole espresso in modo unanime alla Camera, completa un lungo e complesso percorso, iniziato nel 2002 con la Convenzione tra Italia e San Marino, il Protocollo aggiuntivo del 21 marzo, di fatto mai ratificata, modificata il 13 giugno 2012. Questo percorso è andato maturando grazie al consolidamento dei rapporti di amicizia e cooperazione tra le istituzioni dei due Paesi, che quotidianamente si alimenta e rafforza attraverso i comportamenti e gli scambi dei propri cittadini. Credo che il miglior collante per la rinnovata amicizia sia proprio la condivisione di quei principi di legalità e trasparenza che il Partito Democratico

Per favore, prego la Presidenza di fare tutto il possibile per evitare che si commettono reati di qualunque genere, almeno in quest'Aula.

Presidente, onorevoli colleghi, mettere in dubbio, non votandolo, l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche sarebbe incomprensibile. Si tratta di ratificare la firma siglata dai due Paesi a Vilnius il 21 febbraio 2013, che noi invitiamo a votare all'unanimità. Ci troviamo al cospetto di una Nazione relativamente giovane, senza l'incubo dell'Unione Sovietica che, nonostante tutto, non ha lasciato segni della sofferenza passata nella società e nei territori. Un paese, la Lituania, in progressiva crescita, pieno di entusiasmi e di iniziative, per certi versi assai più civile ed in linea con le scommesse contemporanee del nostro Paese. Infatti, mai come ora i due Paesi hanno necessità di rapporti diplomatici

si scontrerebbe con le logiche europeiste e di Unione alle quali si fa riferimento continuamente per il futuro degli Stati Uniti d'Europa. Il mio auspicio personale è che ci si impegni nel far riferimento ad una società come quella lituana, che ha un sistema di servizi di gran lunga più all'avanguardia di quello dell'Italia. effettuati con mezzi nuovi ed efficienti e le linee ferroviarie sono al passo con i tempi. È una Nazione «verde», avvezza già da anni alla raccolta differenziata dei rifiuti e attenta alla conservazione dei grandi palazzi rinascimentali ed al patrimonio artistico-culturale. È una Nazione dalla quale l'Italia può attingere quella serenità del progetto smarrita convulsamente nei vortici delle Nazioni più blasonate ed altrettanto caotiche. Assicurare, come dice il preambolo dell'Accordo: «(...) che le attività delle rispettive rappresentanze diplomatiche siano condotte con la massima dignità e decoro, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche» è una necessità dalla quale non si potrà prescindere ed un voto ostile risulterebbe immotivato e dannoso. Per questi motivi chiedo il voto favorevole all'Accordo e anche di

dato dalla Lituania, al pari di altre Repubbliche uscite dal giogo sovietico negli ultimi anni, quello di sapersi modernizzare e di

ci piace il concetto di integrità e di buona conservazione presente nell'articolo 3; ci piace l'idea del riconoscimento del carattere storico e artistico e l'impegno, nella riqualificazione di questo stabile, a rispettare la normativa sulla conservazione dei beni culturali. Nella dichiarazione di voto, che per il Movimento 5 Stelle è favorevole, permettetemi per un momento di ribaltare la questione, senza che sembri un *off topic*. Il tema del patrimonio immobiliare pubblico del nostro Paese è stato più volte all'ordine del giorno: conosciamo bene l'importanza per le casse dello Stato della dismissione del patrimonio pubblico inutilizzato; sappiamo anche che, in un momento di forte crisi economica, che obbliga i Governi a chiedere sacrifici sempre maggiori ai cittadini, risulta sicuramente prioritaria la lotta agli sprechi e la riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Ci troviamo davanti ad un Paese, la Lituania, che decide di investire in un bene storico, un bene che rappresenta

abbiamo anche noi all'estero) di proprietà dello Stato italiano, verificandone il reale utilizzo, distinguendo quali immobili siano veramente necessari all'attività di rappresentanza e quali siano solamente un costo e pertanto vadano dismessi. Come Movimento 5 Stelle riteniamo che non sia sensato dismettere immobili laddove, poi, questo implichi la necessità di provvedere contestualmente all'affitto di un altro immobile al fine di garantire le funzioni di degna rappresentanza della nostra cultura, della nostra storia, del nostro *made in Italy*. Ci sembra altrettanto importante non acquisire immobili laddove siano presenti immobili sottoutilizzati, che sarebbe opportuno - come sta facendo la Lituania - recuperare e riqualificare.

di ottemperare agli Accordi internazionali. Per questo motivo, dichiariamo il nostro voto favorevole e auspichiamo che il Governo italiano e lo Stato italiano possano muoversi in una simile direzione.

che non significa mettere in discussione quanto andremo a votare, perché voteremo favorevolmente e, anche noi, daremo il nostro assenso. Nell'articolo 1

il Governo della Repubblica di Lituania faciliterà il Governo della Repubblica italiana, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche

chiedo scusa per la mia riflessione ad alta voce; nel caso in cui non dovesse essere così, sarebbe bene attenzionare prima ancora di andare a votare. Siccome il Gruppo del PdL ha già deciso di esprimere voto favorevole

io intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, con due brevi osservazioni. La prima è che, anche se non sarà stata del tutto pertinente con l'ordine del giorno, io condivido l'osservazione della senatrice Mussini sulla esigenza di razionalizzare la nostra presenza a livello internazionale, anche dal punto di vista degli immobili. Questa è una annosa questione, che dovrebbe entrare pienamente nella famosa *spending review* del Ministero degli affari Naturalmente questo comporta, o dovrebbe comportare, la definizione di un rapporto diverso con il Ministero dell'economia e delle finanze, perché oggi, qualunque eventuale cessione, vendita, alienazione dei nostri immobili all'estero, anche quelli non pienamente utilizzati, finirebbe nel calderone del demanio e il ricavato non potrebbe essere riutilizzato per per acquisire nuove sede in situazioni nuove, in Paesi oggi più interessanti dal punto di vista diplomatico. È necessario prendere in mano questa questione. Non è un tema nuovo: noi abbiamo provato a spingere nella scorsa legislatura, continueremo a farlo,

all'articolo 3 si dice: «Il Governo della Repubblica di Lituania si impegna ad eseguire a proprie spese i necessari lavori di rinnovazione dell'immobile che lo stato attuale richiede ed a mantenere a sue spese l'immobile nella sua integrità ed in stato di buona conservazione. buona conservazione. Considerato il carattere storico e artistico dell'immobile (...)». In sostanza, il punto è che noi abbiamo un immobile di pregio, in condizioni evidentemente fatiscenti; lo offriamo a titolo gratuito alla Lituania per poter ospitare la sua rappresentanza diplomatica, in cambio di lavori che, in questo modo, valorizzano un immobile

in ordine a una modalità molto singolare di rimpatrio forzato della moglie del dissidente kazako, la signora Alma Shalabayeva, perché credo che questo lo richieda l'opinione pubblica del nostro Paese. Qualsiasi eventuale reato o comportamento, anche da condannare, non può giustificare sul territorio nazionale una pratica del tutto ignara delle regole e anche delle garanzie che vengono date ai cittadini che sono nel territorio nazionale e che eventualmente facciano richiesta di asilo politico. Questa è una vicenda che non può passare sotto silenzio e su cui noi non accettiamo lo scaricabarile tra l'uno e l'altro componente del Governo. L'Esecutivo ha una responsabilità collegiale e collegialmente ci deve dare una risposta. Scusi, signor Presidente, ma volevo integrare le cose che sono state dette, perché è assolutamente necessario.

Signor Presidente, signora Vice Ministro, colleghi, proverò brevemente a descrivere alcuni motivi di sicuro interesse della Convenzione, la cui ratifica ed esecuzione siamo chiamati ad autorizzare questa sera.

si propone l'obiettivo di promuovere condizioni di vita e di lavoro più dignitose per la gente di mare, oltre che condizioni più eque di concorrenza per gli operatori e i proprietari delle navi. Si tratta di una Convenzione «consolidata» perché contiene un insieme di *global standards*, che figurano in 68 Convenzioni o raccomandazioni in materia di lavoro marittimo adottate dall'OIL dal 1920 ad oggi. È interessante ricordare che tra le organizzazioni internazionali l'OIL è infatti una di quelle dotate di maggiore storia e lignaggio. L'atto costitutivo dell'Organizzazione fu redatto da una Commissione internazionale del lavoro, istituita addirittura dal Trattato di Versailles, quello con cui si concluse la prima guerra mondiale. Da allora il numero dei Paesi membri è cresciuto fino a raggiungere 177 Stati. Voglio ancora ricordare e sottolineare che, fin dalle sue origini, l'OIL ha la particolarità di avere una struttura «tripartita»: è cioè composta non solo dai rappresentanti dei Governi, ma anche dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro di ciascun Paese, che possono così discutere, a livello globale, delle esperienze e delle politiche nazionali. Alla Conferenza internazionale del lavoro, che si svolge una volta l'anno, ogni Stato è rappresentato infatti da quattro delegati: due del Governo, uno per i sindacati e uno per gli imprenditori. Con atti normativi come quello oggi all'esame dell'Assemblea, l'Organizzazione internazionale del lavoro svolge un lavoro prezioso: da un lato promuove condizioni di vita e di lavoro più dignitose per i lavoratori di tutto il mondo, indipendentemente dal Paese in cui si trovano e in cui svolgono la propria prestazione, dall'altro garantisce migliori condizioni di concorrenza tra gli operatori economici. Lo sappiamo tutti: fissare regole internazionali che valgono per tutti è infatti l'unica strada per porre un freno a quel *dumping* sociale, a quella straordinaria differenza tra le condizioni di lavoro nel Nord e nel Sud del mondo, tra i Paesi più ricchi e quelli emergenti, che distorce l'economia mondiale e causa ogni giorno tragedie piccole e grandi. Proprio per questo l'OIL è generalmente riconosciuta come una delle esperienze di maggior successo tra le organizzazioni internazionali. Nella sua attività, pur con tutte le difficoltà e tutti i suoi limiti, tale organizzazione riesce spesso a dare un contributo reale a quel «governo della globalizzazione» che tante volte viene invocato come unico modo per conciliare l'apertura dei mercati e delle economie con il rispetto dei diritti umani e della concorrenza. Sul merito voglio richiamare l'organizzazione dell'Aula solo sul fatto che le Commissioni riunite durante l'esame hanno convenuto di sopprimere l'articolo 4 recante la normativa da applicarsi ai lavoratori extracomunitari non residenti nell'Unione europea. Il testo originario del disegno di legge prevedeva, all'articolo 4, che a tale rapporto fosse applicabile la legge regolatrice del contratto di arruolamento, in analogia a quanto disposto per i marittimi italiani e comunitari. Sopprimendo tale articolo, si è mantenuta quindi in vigore la normativa attuale, che prevede che il rapporto di lavoro in questione rimanga regolato dalla legge scelta dalle parti. Tale emendamento è stato frutto di un esame approfondito, di un'analisi della legislazione comparata dei principali Paesi europei e di un confronto con i sindacati, che hanno espresso il loro favore per tale modifica. L'approvazione dell'emendamento non diminuisce quindi le garanzie nei confronti dei lavoratori marittimi, che già trovano altre forme di tutela, ma evita la perdita di competitività della marina mercantile italiana. Mi soffermo, infine, sull'orizzonte temporale entro cui dovremmo realizzare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione. Il 20 agosto 2012 sono stati infatti raggiunti i presupposti per l'entrata in vigore della Convenzione, che erano presupposti «misti», ossia riferiti sia al numero di Stati che alla quota della flotta mercantile mondiale. Con le ratifiche delle Filippine e della Russia si sono raggiunte, da un lato, le trenta ratifiche e, dall'altro, la soglia del 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale. La Convenzione entrerà dunque in vigore a dodici mesi da quella data.

È infatti essenziale che, entro quella data, gli armatori italiani possano ottenere dall'amministrazione italiana competente, cioè dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le certificazioni che attestino che le proprie navi sono conformi ai requisiti posti dalla normativa in vigore, sul piano internazionale, in tema di sicurezza e di condizioni di lavoro a bordo. La mancata ratifica entro quel termine, infatti, esporrebbe il settore armatoriale ed i lavoratori agli effetti negativi di una significativa perdita di competitività del nostro Paese. Le navi battenti bandiera italiana prive di certificazione potrebbero addirittura essere sottoposte al rischio di provvedimenti di fermo amministrativo da parte delle autorità dei Paesi di scalo che hanno ratificato la Convenzione. ratificato la Convenzione. Considerato che il mercato globale del trasporto marittimo risente di per sé, fortemente, delle difformità nelle regole applicabili da parte delle autorità di regolazione in ciascun Paese, a fronte di questo rischio gli operatori delle attività di commercio internazionale potrebbero considerare preferibile orientarsi su vettori di altri Stati. colleghi, il disegno di legge in esame reca al Capo I, all'articolo 1, l'autorizzazione alla ratifica e, all'articolo 2, l'ordine di esecuzione. Al Capo II reca invece le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione oggetto di ratifica. Gli interventi in questione sono volti a soddisfare le esigenze evidenziate dal Comitato europeo dei diritti sociali e la richiesta di modifica avanzata dalla Commissione di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni OIL. Nel merito, essi adeguano le disposizioni del codice della navigazione, introdotte nel nostro ordinamento nel contesto socioeconomico del 1942, e che risultano in contrasto con il portato dei principi giuridici attuali, rendendo effettive le modalità di tutela dei diritti dei lavoratori a bordo delle navi. In particolare, l'articolo 3 apporta alcune modifiche al codice della navigazione. Il comma 1 novella l'articolo 368 del codice, al fine di prevedere che la disciplina del rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane, di cui al Libro II, Titolo IV, Capo V del Codice, trovi sempre applicazione e non, come attualmente previsto, solo a condizione di reciprocità (ossia a condizione che lo Stato di cui lo straniero arruolato è cittadino assicuri eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la sua bandiera). I commi 2 e 3 del medesimo articolo novellano gli articoli 1091 e 1094 del codice, che prevedono i delitti, rispettivamente, di diserzione e di inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio, circoscrivendo l'ambito di applicazione della sanzione penale alle sole condotte che cagionino un pericolo per la vita e l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della navigazione. Nei casi in cui, invece, non si configuri una violazione dei suddetti beni primari e le condotte siano esclusivamente lesive dell'efficienza e del buon andamento dell'organizzazione di bordo, la sanzione penale viene sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria. Come è stato anticipato dal collega relatore Russo, le Commissioni riunite hanno previsto la soppressione dell'articolo 4 del disegno di legge, che modifica la legge applicabile al rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale. L'articolo 4 del testo proposto dalle Commissioni riunite aumenta da quindici a sedici anni l'età minima richiesta per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare. L'articolo 5 reca modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi e assistenza sanitaria a bordo. Mentre attualmente il certificato medico attestante l'idoneità dei marittimi a lavorare a bordo delle navi ha sempre durata di due anni dalla data del rilascio, il comma 1, pur conservando in via generale il suddetto termine di durata di due anni, lo riduce a un anno per i marittimi che hanno meno di diciotto Inoltre, con decreto ministeriale può essere previsto un periodo di validità più breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo. Sempre a un decreto ministeriale è rimessa la disciplina dei casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza ovvero se il periodo di validità del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore a tre mesi. Ai sensi del comma 2, le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria. L'articolo 6 abroga l'articolo 36 della legge n. 1045 del 1939, recante disposizioni applicabili ai marittimi di colore, incompatibili con l'impianto costituzionale. L'articolo 7 reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle spese di missione connesse alla partecipazione di rappresentanti designati dal Governo alle riunioni del Comitato tripartito speciale, avente la funzione di seguire permanentemente l'applicazione della Convenzione, ai sensi dell'articolo XIII della Convenzione stessa. *(Applausi dei

Signor Presidente, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle annuncio il voto favorevole alla ratifica Lo dico per sgombrare il campo da ogni dubbio e, tuttavia, non rinuncio, a titolo personale e a nome degli amici cittadini a cinque stelle, a rimarcare alcune considerazioni che sono già emerse nel dibattito. La Convenzione è indubbiamente un passo avanti, e questo lo abbiamo appreso ascoltando le associazioni di categoria ed i lavoratori. La certificazione del lavoro marittimo sulle condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi è un progresso verso la omogeneizzazione ed il miglioramento della condizione dei lavoratori imbarcati di ogni nazionalità. Purtroppo, saranno i singoli Stati a rilasciare detta certificazione e qualcuno potrebbe decidere di diminuire un po' il numero e la qualità dei controlli, pur di accaparrarsi il favore di certi armatori, poco interessati alla propria reputazione. Tuttavia, vogliamo essere ottimisti; un detto popolare recita: «L'ottimo è nemico del buono». Oggi, quindi, ratifichiamo una buona normativa; il tempo ci dirà se sia perfettibile e se darà buoni frutti. Infine, permettetemi di salutare con sollievo e un pizzico di compassione, per chi questa legge l'aveva redatta e approvata, l'abrogazione dell'articolo 36 della legge n. 1045 del 1939, che stabiliva un regime di separazione rigido sulle navi per le persone di colore.

spesso usiamo questo spazio per commemorare qualcuno o per riportare all'attenzione dell'Aula un evento tragico. Io invece oggi voglio condividere con voi una bella notizia e contemporaneamente lanciare un appello. Marianna è una bambina di nove anni seguita presso il reparto di oncologia pediatrica della Seconda Università degli studi di Napoli. A sei anni, con un apparente, banale e comune episodio febbrile, comincia il suo calvario: leucemia linfoblastica acuta. due anni di estenuanti cure per debellare il male, sembra guarita. Ma si tratta di un solo mese di calma apparente. Ritorna il male: in gergo si chiama recidiva. I medici comunicano alla madre che la sola cura per la piccola Marianna è il trapianto di midollo osseo. Serve dunque un donatore (questo a dicembre 2012). Marianna aspetta, pur rischiando la vita ogni giorno. Non può fare altro che aspettare e sperare. Molte volte le famiglie aspettano inutilmente, impotenti, perché non sempre i piccoli pazienti ammalati di patologie onco-ematologiche hanno in famiglia un fratello compatibile. Alla fine però arriva anche per Marianna una possibilità, una speranza: un donatore compatibile. Ad inizio luglio 2013 la possibilità di avere una vita normale sembra riprendere forma. Le statistiche dicono che la possibilità di trovare un donatore compatibile è di 1 su 100.000. Il mio appello è dare maggiore attenzione alla donazione del midollo osseo. Occorre attivare una capillare azione di informazione, perché purtroppo in Italia molti non sanno della grande possibilità di combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali contenute nel cordone ombelicale. In Italia in pochi sanno che donare il midollo osseo è una procedura semplicissima: per iscriversi al Registro mondiale dei donatori, e quindi per entrare nel *database*, basta un semplicissimo prelievo di sangue. La donazione vera, se si è chiamati a salvare la vita di qualcuno, può essere fatta con un metodo classico, ossia il prelievo delle cellule staminali dalla cresta iliaca, eseguito in anestesia (quindi senza dolore per il donatore), un metodo innovativo, che consiste nel prelievo delle cellule staminali da sangue periferico (con una semplice donazione di sangue, per intenderci), dopo aver assunto nei tre giorni precedenti la donazione un farmaco, privo di effetti collaterali per il donatore. Si pratica dunque una banale trasfusione di sangue e si salva una vita. Voglio ricordare inoltre che in questo periodo tutti i centri trasfusionali d'Italia sono in emergenza. Purtroppo, durante il periodo estivo, il numero dei donatori di sangue diminuisce drasticamente; di contro, invece, aumenta il numero dei pazienti che necessita di trasfusioni periodiche. Il mio appello è di ricordare a tutti che la donazione del sangue dovrebbe essere un dovere civico più che un atto di elitaria generosità ed umanità. Peccato che tutti siamo sempre troppo impegnati a pensare ad altro, perché in fondo «il problema è di chi c'è l'ha». Per una volta pensiamo a chi sta male, a chi aspetta, a chi ha bisogno di una mano, con i fatti e non solo con belle ed inutili parole. Salvare una vita è più semplice di quanto si pensi.

«Storie che interrogano. Quelle che quotidianamente segnano il territorio della Valle di Susa, terra d'acqua e di roccia, terra di innumerevoli bellezze nascoste tra boschi e sentieri e deturpate da quel nuovo che avanza e che copre tutto d'asfalto e di cemento. E che da alcuni anni avanza con recinzioni, fili spinati (i migliori), le concertine, patrimonio di altre terre, quelle di Gaza, ad esempio. Le vicende narrate intorno a quest'opera dell'alta velocità, a questo primo minuscolo inizio di galleria geognostica, sono quelle che regolarmente riempiono le pagine dei giornali: violenze, lanci di sassi, resistenze... peccato che non si parli mai di quei terribili lacrimogeni al CS, vietati in guerra ma utilizzati qui come in altre piazze, gas cancerogeni e mutageni... Storie vere e storie costruite si confondono in questo non luogo della democrazia, dove coloro che giungono vengono fotografati, filmati, identificati e pazienza se la Costituzione afferma che i cittadini sono liberi di circolare su tutto il territorio nazionale. Insomma, ovunque, ma non qui. Ultimamente si sentono anche tante storie sulla grande opera del TAV: ci sono strani incidenti, mezzi che si incendiano, operai che vanno al pronto soccorso. Tante storie da verificare, ma regolarmente assegnate alla violenza scatenata dai "no TAV". L'ultima storia è quella dell'inizio della scorsa settimana, quando di notte a due mezzi del cantiere è stato appiccato fuoco alle gomme, con dei cubetti di "diavolina", quelli utilizzati per accendere le stufe. Un principio d'incendio prontamente spento da alcuni operai che sono intervenuti (quindi erano lì!). Questa la storia uscita sui giornali, che naturalmente non ha mancato di nominare i soliti "no TAV" come probabili esecutori. Ma accanto a questa storia ci sono altri dettagli. Nel pomeriggio precedente un amministratore dell'alta valle aveva affermato che la sera sicuramente ci sarebbe stato qualche nuovo tafferuglio. Ma l'unica cosa in programma, e poi avvenuta regolarmente, erano la cena con i balli occitani e poi il finale con il falò. Poi tutti a nanna. Immaginarsi la sorpresa nell'apprendere del principio d'incendio il giorno dopo... La domanda allora è inevitabile: chi e perché aveva in mano il cerino? Perché circolava la voce che qualcosa sarebbe accaduto? In questa direzione sarebbe opportuno cercare risposte, evitando così di trovare più facili soluzioni a portata di mano. E cercando, anche se questo è molto più impegnativo e faticoso, di ascoltare le ragioni di una popolazione che sta parlando a muri di gomma e che vorrebbe ritrovare la possibilità di dialogare tra persone aventi gli stessi basilari desideri e gli stessi diritti. Gabriella Tittonel, valsusina».

Grazie Massimo Caleo, che è intervenuto per primo su questi eventi sismici, fossero costruite bene: infatti non ci sono stati né morti né feriti.

ne sappiamo qualcosa noi di cultura socialista dopo Sigonella. grandi capacità e competenze e forse sarebbe opportuno che il Governo valutasse l'opportunità di sostituirlo per assoluto fallimento, almeno nel contesto del terremoto della Lunigiana e della Garfagnana, proprio perché non si è più visto, ha lasciato le popolazioni a dormire nelle tende e manca qualsiasi notizia e informazione. La cosa più brutta è quella di non avere informazioni, continuando la terra a tremare e continuando i tecnici a girare su se stessi, perché nessuno più si prende la responsabilità nemmeno di fare entrare le persone in chiesa a pregare. Grazie a Dio le scuole sono chiuse, perché altrimenti non avremmo più avuto nessun edificio

ad intervenire presso il Governo, affinché anche quelle terre siano considerate - come ha detto il senatore Giovanardi - alla stregua di tutte le altre terre colpite dai terremoti in Italia.

Grazie